Onorevoli colleghi, comunico che, qualora nella seduta di questa mattina presso la Camera dei deputati non si raggiungesse il *quorum* richiesto per l'elezione di un giudice costituzionale, il Parlamento in seduta comune sarà nuovamente convocato oggi pomeriggio alle ore 16. In tal caso, la seduta della nostra Assemblea avrà inizio alle ore

Commissione antimafia e trattano la materia del grave fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito.

aveva il compito, nell'ambito dell'attività della Commissione antimafia, di esaminare i profili inerenti al riciclaggio. Un intervento del senatore Raffaele Lauro in Commissione antimafia del 13 gennaio 2009, particolarmente incisivo, ha richiamato l'attenzione dell'intera Commissione, e quindi del VI Comitato, sul problema del del gioco lecito ed illecito, con tutte le conseguenze e gli effetti ad esso collegati.

inviato per i profili attinenti le sue competenze (la Commissione Grandi si muoveva nell'ambito di un lavoro della Commissione finanze della Camera).

procedendo a numerose audizioni: il Comitato ha infatti i Monopoli di Stato, la Guardia di finanza, le associazioni antiusura, la Confindustria, la procura nazionale antimafia.

Da questo confronto con i diversi interlocutori si è evidenziato come il settore del gioco costituisca il punto d'incontro di plurime gravi distorsioni dell'assetto socio‑economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani al rischio di erosione, l'interesse del crimine organizzato, la vocazione allo spasmodico arricchimento di taluni concessionari, che operano sovente in regime di quasi monopolio, il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. E soprattutto, emergeva come, nei periodi di crisi economica, tale fenomeno degenerativo si accentui maggiormente in quanto, nella impossibilità di un aumento della tassazione, si implementa il ricorso ad incentivazioni della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento.

in Italia tra il 2003 e il 2010, ossia sette anni, è stata complessivamente di 309 miliardi di euro.

Il settore che ha conosciuto il maggiore incremento, rappresentando cento dell'intera raccolta da gioco, è quello collegato agli apparecchi da intrattenimento. Cresce moltissimo anche il settore del Gratta e Vinci.

con un aumento della raccolta da gioco del 13 per cento, le entrate dell'Erario sono diminuite dello 0,8 È un paradosso spiegato dal fatto che il sistema di tassazione varia da gioco al gioco, nel senso che non è uniforme,

A questo fenomeno si collega un costo sociale elevato.

che invece di migliorare la propria condizione di vita finisce col costituire una vera e propria aggressione dei beni e dei patrimoni delle famiglie, intaccando i portafogli prima ancora della salute dei dei giocatori. È particolarmente allarmante che nel settore che più ha visto la crescita della raccolta, ossia il settore delle macchine da gioco, gli accertamenti fatti negli anni precedenti

alla rete di controllo e, quindi, sfuggivano a qualsiasi forma di tassazione. patologico un particolare aspetto: le macchine da gioco, qualora vengano messe messe fuori mercato perché necessitano interventi di manutenzione o perché si è in attesa dell'autorizzazione,

che addirittura in uno stesso giorno furono immagazzinate in un locale di un paesino della Sicilia ben 27.000 video macchine. La Guardia di finanza, che accertò questo dato, disse che, messe una sopra l'altra, si arrivava all'altezza dell'Etna. Queste macchine risultavano tutte in un magazzino, ossia si creava un magazzino virtuale di macchine che però erano regolarmente in funzione. monopoli di Stato, di fronte a questa situazione, si è mossa seguendo due direttrici: da un lato, creando un portafoglio di gioco più ampio rispetto al passato, onde determinare, di fatto, una sorta di offerta concorrenziale al gioco illegale; dall'altro, apprestando un sistema di controllo e regolarizzazione

rendere la macchina non funzionante se non dotata di una *smart card,* un *microchip* che, collegato al sistema SOGEI dei Monopoli, consentiva la lettura del monte delle giocate che ogni macchina produceva. Questo sistema è stato ritenuto particolarmente efficace, in quanto è in grado di controllare effettivamente quello che veniva incassato dalle diverse macchine. Sistema ermetico: senonché, dagli accertamenti svolti dalla Commissione e dal Comitato e dall'acquisizione della documentazione delle indagini, si è visto che la criminalità

che deviava i dati di raccolta da gioco, trasmettendo al sistema SOGEI (alla rete) cento del totale della raccolta da gioco. L'80 per cento veniva in questo modo sottratto ad una possibile tassazione. Un altro sistema che le indagini citate nella relazione hanno evidenziato era la possibilità studiata di trasformare le macchine

A fianco a questo fenomeno, di interesse per l'enorme quantità di danaro, si sviluppa un

I numeri dei malati da gioco compulsivo hanno superato il milione di unità. Dietro vi è la disperazione, è lo sfruttamento attraverso l'usura, vi è l'interesse della criminalità e la disperazione delle famiglie. È vero, Confindustria ha richiamato l'attenzione dicendo che in fondo la stima del giocato per ogni italiano è pari ad una colazione ogni giorno,

colazioni e chi non ne fa neanche una, e così avviene nel gioco. Si dice anche che poi le vincite sono distribuite, ma si è accertato che chi vince reinveste nel gioco,

di maggiore raccolta da gioco, specialmente nel settore del Gratta e Vinci, sono quelli di riscossione della pensione. È la povera gente che viene sollecitata continuamente e stimolata nella speranza della vincita.

quale ha evidenziato un dato allarmante: il gioco, comprese le scommesse su eventi sportivi, per i notevoli introiti che vengono assicurati a fronte di rischi giudiziari relativamente contenuti, è ormai diventato la nuova frontiera della criminalità organizzata di tipo mafioso.

(oltre 70 miliardi di euro l'anno), vi è un settore del gioco illecito che sfugge totalmente ai controlli, che è stimato dalla Guardia di finanza essere pari a tre volte il monte della raccolta lecita. I fenomeni sociali sono di grande evidenza, così come i fenomeni criminali collegati al gioco e alla disperazione del cittadino che cerca la vincita,

l'offerta dei *videopoker* accessibili a tutti, senza possibilità di ancorare forme di controllo deve vincere il principio del diritto di stabilimento, nel senso che chiunque può svolgere questa attività. In Commissione antimafia

esteri. Il complesso di queste ragioni, che ho cercato di sintetizzare in questi pochi minuti - ma la relazione contiene dati, è molto ampia ed è articolata per capitoli - ha suggerito alla Commissione di sollecitare il Parlamento e l'Aula ad una riflessione che possa portare ad una inversione di tendenza, considerando che in Italia soltanto nel settore dei videogiochi esiste

400.000, ripeto: le troviamo ovunque. Tutto questo è controllato in buona parte dalla criminalità, che impone il controllo del territorio attraverso i gestori, e si traduce in un disastro per i giovani, per gli anziani, per le famiglie. Affidiamo alla vostra valutazione,

è stato pubblicato sul bollettino del Ministero dell'economia e delle finanze un dato secondo cui nel primo quadrimestre del 2011 le entrate totali relative ai giochi, incluse le imposte classificate come dirette e indirette, sono risultate di 4.730 milioni di euro, con una crescita rispetto al primo quadrimestre dell'anno precedente del 19,6 per cento, ossia 774 milioni di euro in più. Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività di gioco è di 4.535 milioni di euro: più 775 milioni, pari al 20,6 per In questi quattro mesi, si legge sempre nel bollettino, hanno contribuito in maniera particolare alla crescita delle entrate erariali relative ai giochi i proventi del gioco del lotto, che sono stati pari a 2.278 milioni di euro. Questi dati, paragonati allo stesso periodo di riferimento del 2010, segnano una crescita di quasi 671 milioni di euro, 41,8 per cento. Per quanto riguarda invece i proventi degli apparecchi da intrattenimento e i congegni di gioco,

dell'incentivo al gioco tramite la pubblicità fatta da uno Stato biscazziere - ripeto, uno Stato biscazziere - che incita al gioco soprattutto i

al senatore Li Gotti, al senatore Lauro e al presidente Pisanu per questa inchiesta sulle infiltrazioni criminali nel mondo del gioco.

non solo per i biscazzieri ma anche per la criminalità organizzata. La pubblicità dilagante incentiva il poker *on line*,

le grandi banche, le agenzie di *rating -* quelle che ieri hanno declassato l'Italia, come Moody's e Standard & Poor's - e i grandi banchieri d'affari hanno invitato i cittadini ad indebitarsi. La nuova ideologia è quella del debito: non più quella della produzione, ma quella della finanza e del gioco d'azzardo. Non esistono più i valori

si gioca, si reinveste e, se si vince qualcosa con il Gratta e Vinci, si apre una spirale che porta alla ludopatia. La pubblicità dilagante incentiva il poker *on line* e altri giochi d'azzardo e a caderne vittime, perdendo soldi, sono anche i minorenni, anche i ragazzi che nel gioco investono la paghetta.

risultano coinvolte circa un milione di persone come avventori, e sono stime approssimate per difetto. E questa filiera del gioco legale comprende l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, i concessionari, i gestori, gli esercenti, e così via. E l'amministrazione fornisce ai concessionari il benestare all'operatività che questi espletano attraverso gli esercenti. Si è parlato di tutte queste macchinette «mangia soldi» e «rovina-famiglie»,

- il comunicato stampa del senatore Lauro. Anche lui è impegnato a riportare la legalità nel gioco, dove (prima l'avevo ricordato a memoria, e adesso leggo) «l'Italia sta diventando la Bengodi europea del gioco, una fabbrica di illusioni e di disperazione che, come un cancro, divora quotidianamente i redditi delle famiglie italiane,

quella dell'economia reale, è fatta di sacrifici, di impegno, soprattutto per i giovani, di studio, e soprattutto di sobrietà, di non illudere il prossimo. Ripeto: noi avevamo approvato quelle mozioni al Senato non molto tempo fa fa ed il fenomeno del gioco d'azzardo è diventato un fenomeno in forte espansione, anche per l'ausilio di nuove modalità telematiche Internet - che ne hanno consentito l'accesso ad un pubblico sempre più ampio. E chi sono quelli che utilizzano Internet? Anche quelli della mia generazione, è vero, ma sono soprattutto i giovani, che fanno le partite di poker *on line* e si giocano non solo la paghetta e si indebitano in un vortice che non si sa dove porta, se non a rovinare le famiglie. Voglio altri, un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel quale si dice che ci sono circa un milione e mezzo di adulti a rischio di ludopatia. Mi accingo

«È chiaro l'intento del Governo liberale e liberista: tassare la speranza in un momento in cui questa è vista dal giocatore come l'unica via d'uscita da una condizione insopportabile; il tutto senza tenere in considerazione le ricadute sociali». E concludeva: «Dopo tre anni di non governo è arrivata la prima liberalizzazione epocale: potremmo giocare di più da casa e con poste più alte; i datori di lavoro potranno offrire il Gratta e Vinci in busta-paga hold'em al posto della tredicesima. Il ministro Brunetta potrà organizzare estrazioni ai tornelli, Nitto Palma farà giocare i detenuti e La Russa offrirà licenze premio collegate al Superenalotto». Signora Presidente, uno Stato serio non propaganda, non incentiva il gioco e non fa lo Stato biscazziere, ma tutela i propri cittadini. È questo che noi ci aspettiamo da questo Governo. Ringrazio ancora una volta la Commissione antimafia per l'egregio lavoro che ha voluto fare.

questo Parlamento - tanto e troppo vituperato negli ultimi tempi - abbia deciso di occuparsi di un problema gravissimo come quello del gioco e, in particolare,

del senatore Li Gotti, che tutti abbiamo condiviso. Devo anche dire con grande soddisfazione che in Commissione antimafia si lavora quasi sempre all'unanimità

e a dimostrazione del fatto che su un tema così importante per il nostro Paese è stata possibile una convergenza che credo faccia onore a tutti i colleghi. Il senatore Lauro ha ripescato la Commissione Grandi che era andata a morire perché andava a morire quella legislatura.

è dal nostro Paese e dal nostro Stato incentivato quotidianamente e, come diceva il senatore Lannutti, non si può pensare ad uno Stato biscazziere. Non illudiamoci: il gioco porta all'erario tanta moneta, e quindi pensare che non si debba più giocare o autorizzare il gioco mi sembra illusorio e, talvolta, anche controproducente;

e a muovere le acque su questo tema, perché la malavita e la criminalità organizzata entrano negli appalti, la criminalità organizzata entrano negli appalti, nell'acquisto di beni immobili e di esercizi pubblici; la criminalità organizzata entra là dove c'è la moneta. Nel gioco d'azzardo c'è tanta moneta, e quindi è impensabile che la criminalità organizzata, si chiami essa mafia, camorra o 'ndrangheta, si astenga da questo settore. Se questo è vero, la necessità di paletti è urgente, perché il gioco, sia esso autorizzato o illecito - è addirittura banale sottolinearlo - porta a suicidi,

paletti devono riguardare soprattutto i minori, poiché la normativa è poca cosa oggi

Mi fa piacere che si sia pensato alla tracciabilità del denaro, per cui chi gioca 1.000 euro deve essere identificato: un'identificazione seria, un'identificazione seria, che deve riguardare anche coloro che giocano *on line*. Mi fa piacere anche pensare che per il rilascio dell'autorizzazione sia necessaria la certificazione antimafia (tanto bistrattata da questo Governo, in particolare dal ministro Brunetta, che la ritiene inutile) e l'istituzione di un registro dove poter segnalare e segnare ogni cosa che riguarda il gioco. Il gioco illecito in particolare porta a reati gravissimi, all'usura, all'evasione fiscale.

a dilatare le risorse della criminalità organizzata. È bene che si metta un freno a questo fenomeno, ed è bene che ci sia l'attenzione di tutto il Parlamento, del Senato e della Camera.

approvate dalla Commissione antimafia nelle sedute del 17 novembre 2010 e del 20 luglio 2011, approvazione, voglio sottolinearlo, avvenuta all'unanimità. l'odierno dibattito è la continuazione di quello avvenuto il 29 giugno 2011 in Senato, quando sono state discusse e approvate sei mozioni sul gioco d'azzardo presentate da tutti i Gruppi politici.

condividere e drammaticamente evidenziano come il settore del gioco rappresenti il punto di convergenza di numerose, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico del nostro Paese: l'interesse del crimine organizzato ed il proliferare di fenomeni criminali connessi come usura, estorsione, riciclaggio; il rischio di erosione dei redditi degli italiani; l'interesse all'arricchimento di taluni concessionari che operano, spesso, in regime di quasi monopolio; la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Soprattutto emerge come nei periodi di crisi economica il fenomeno degenerativo del gioco si accentui: non potendosi aumentare la tassazione, si implementa il ricorso ad incentivazioni della "malattia del gioco", un meccanismo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento. Nelle conclusioni, le relazioni propongono due iniziative normative assolutamente condivisibili. È già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto cosa è l'industria dei giochi e delle scommesse e che cosa registra. delle scommesse ha registrato negli ultimi anni una rapidissima espansione, sia attraverso la rete fìsica sia a distanza, con una raccolta complessiva aumentata da 15 miliardi di euro del 2003 a 61,4 miliardi del 2010 (il 4 per cento circa del PIL); il tutto generando anche un grosso introito per le casse dell'erario se solo si considera che le corrispondenti entrate erariali si sono attestate a 9,9 miliardi di euro (9,4 miliardi nel 2009).

Se questo *trend* sarà confermato, potremmo avere una raccolta per l'anno in corso che alla fine risulterà superiore ai 72 miliardi. A fronte di questi dati, l'Associazione contribuenti italiani, presentando in questi giorni lo studio «Fisco e Giochi d'azzardo: il triste primato italiano», ha affermato: «L'Italia ha il primato, in Europa, per la maggior cifra giocata ai tavoli da gioco: una media di quasi 2.205 euro a persona, che vengono sottratti all'economia reale, minorenni inclusi, il cui numero è passato da 860.000 unità a 3,2 milioni». milioni». Il rapporto aggiunge poi che «L'Erario si preoccupa più di fare cassa che di sensibilizzare sulle tematiche di dipendenza da gioco». Vorrei a questo punto soffermarmi sulla legislazione e porre una domanda: è vero che la nostra legislazione presenta tali caratteristiche e che pur dopo l'approvazione delle mozioni a fine giugno nulla è stato fatto? Esaminiamo i provvedimenti adottati al riguardo. Per meglio inquadrare la problematica, va ricordato che la legge di stabilità per l'anno 2011 aveva lodevolmente previsto «linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia

contraddittorio) che «per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sarebbero state introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi». Questo secondo progetto è andato avanti combinandosi con altre disposizioni adottate in materia di giochi. Difatti, dopo un periodo di sperimentazione previsto dal decreto-legge a sostegno delle zone terremotate), dal 18 luglio 2011 è possibile giocare a poker con la modalità *cash* che, rispetto a quella del torneo, prevede che si giochi con soldi veri e puntate che vanno da un minimo di 50 centesimi a un massimo di 1.000 euro. Secondo le stime degli operatori, a regime il nuovo gioco dovrebbe produrre un A questo punto è intervenuta la manovra economica, (decreto-legge n. 98 del 2011) che ha previsto all'articolo 24 misure di contrasto al gioco illegale che, non vi è dubbio, tendono a rafforzare il presidio del gioco pubblico che si regge sul sistema concessorio. È stato rafforzato il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincite di denaro per i minori di diciotto diciotto anni (si reintroducono, peraltro, sanzioni che lo stesso Governo aveva diminuito con la finanziaria 2010), si è inteso contrastare i fenomeni di diffusione dei giochi irregolari o illegali, nonché l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio con la previsione dell'obbligo, per le società emittenti carte di credito, per gli operatori bancari, finanziari e postali, di segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti i giochi, le scommesse o i concorsi pronostici con la stessa manovra economica il Governo ha introdotto nuove proposte di gioco d'azzardo. Si può affermare, purtroppo, che il decreto di luglio legalizza il gioco d'azzardo *on line* senza alcuna limitazione di gioco e inserisce nuove possibilità di gioco che possono che possono fondatamente comportare dipendenze. Ha così introdotto il gioco del Bingo a distanza; ha previsto l'apertura di ben 1.000 sale da gioco nelle quali si faranno i tornei di poker dal vivo; è stata data la possibilità di aumentare il numero delle *VideoLottery* fino al 14 cento; si danno disposizioni per l'apertura di 7.000 nuovi punti vendita di scommesse ippiche e sportive. E con la manovra aggiuntiva di agosto il gioco viene ulteriormente incentivato per battere cassa. il decreto-legge n. 138 del 2011, all'articolo 2, attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici, dirette ad assicurare maggiori entrate con un aumento del numero dei dipendenti da gioco d'azzardo. dal dicembre 2010 ad oggi, purtroppo a livello nazionale non vi è stata alcuna novità positiva rilevante. Il Governo si è espresso più volte tramite il sottosegretario che anche nel dibattito avvenuto in Senato nel giugno 2011 ha annunciato che sarebbe stata presentata una proposta di legge-quadro di revisione del comparto del gioco d'azzardo che avrebbe previsto anche interventi sulla ludopatia; in realtà,

occorre tenere conto della contiguità tra gioco legale e gioco clandestino, approvare misure urgenti tese a prevenire e reprimere il gioco d'azzardo illegale, a regolare in modo più rigoroso quello legale, a garantire la trasparenza delle concessioni, ad adottare misure di controllo sui giochi telematici, ad introdurre misure più stringenti a tutela dei minori, a vietare la pubblicità ingannevole e ad impedire il riciclaggio del denaro sporco attraverso le scommesse. Occorre inoltre una pronta riforma strutturale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accompagnata da quella del sistema sanzionatorio e del sistema di verifica. Le relazioni, che oggi approveremo mi auguro all'unanimità,

credo sia davvero una buona scelta politica quella di procedere ad una indagine sul settore dei giochi al fine di individuare proposte normative per contrastare un fenomeno che desta grande allarme sociale, anche per la

antimafia ha il merito di offrire una fotografia aggiornata ed esaustiva sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito. È una rappresentazione che mi permetto di definire agghiacciante, di una società che presenta aspetti gravi e patologici. Il ricorso al gioco è continuamente in aumento ed inoltre emerge la figura di uno Stato connivente. Siamo passati da una situazione nella quale il paradigma dello Stato era autorizzare alcune forme per contenere un comportamento, una condotta di consumo ritenuta un disvalore. Oggi, invece, il modello proposto è quello di una sorta di azione di *marketing*: introdurre nuovi giochi per essere accattivanti e soprattutto per interessare nuove fasce di popolazione. È cambiato l'atteggiamento dello Stato e la relazione sue conclusioni offrono un'agenda di lavoro per fronteggiare l'illiceità e le infiltrazioni mafiose nel settore dei giochi.

«Mi invase una terribile sete di rischio. Forse, passando attraverso tante sensazioni, l'animo non se ne sazia, ma eccitato da esse, ne chiede sempre altre, sempre più intense, fino alla totale estenuazione (...) ero come in preda alla febbre; spostai quel mucchio di denaro sul rosso e ad un tratto tornai in me! Con orrore sentii e compresi immediatamente che cosa avrebbe significato ora per me perdere»; e poi continua: «era in gioco tutta la mia vita!». Sono queste parole che ci fanno capire cosa serve ed è ben contenuto nella relazione. Nella consapevolezza della gravità del fenomeno, si prevede la necessità di armonizzare ai principi europei il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare l'articolo 88 che disciplina

più pesanti a carico degli esercenti che contravvengono alle regole, di misure volte alla tracciabilità dei flussi di gioco e con l'istituzione di un registro delle scommesse. Ottime proposte, che speriamo diventino legge nel più breve tempo possibile. Mi permetto però di segnalare due aspetti, che secondo me vanno non dico inseriti, ma posti alla nostra attenzione: da una parte il tema delle ludopatie (è contenuta un'analisi delle ludopatie, però serve scrivere in modo chiaro, senza se e senza ma, che devono essere inserite nei livelli essenziali di assistenza, e quindi come tali riconosciute come patologie); vorrei porre l'attenzione sulle imposizioni fiscali in materia di giochi. Si tratta di due aspetti che, a mio avviso, ben rientrano nel tema oggetto di discussione, perché il *gambling* patologico e un sistema impositivo ad aliquote variabili

è stato sottolineato anche dal professor Fiasco, che la Commissione antimafia ha audito. Lui dice: «Il gioco d'azzardo patologico è un quadro clinico tipizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità ed è incluso nel manuale statistico diagnostico dei disturbi psichici». È in discussione presso la Commissione sanità un disegno di legge (relatore il senatore Gustavino) del quale credo che dobbiamo chiedere l'immediata calendarizzazione. Continua il professor Fiasco: «La dipendenza dal gioco d'azzardo è un fenomeno reale e riconosciuto in molti Paesi, ma ma non nel nostro». Vi è, dunque, un vuoto di tutela che dobbiamo colmare, per dimostrare alle circa 700.000 persone vittime in Italia del gioco patologico (cui si aggiungono circa 7 milioni di soggetti considerati a rischio) la doverosa vicinanza delle istituzioni, di quelle stesse istituzioni che prima varano provvedimenti che incrementano l'offerta dei giochi e poi si disinteressano delle loro sorti, noncuranti dei disagi sociali ed economici ad essi connessi; ma anche per sferzare un duro colpo alle associazioni criminali sempre più allettate dal comparto dei giochi perché, come ha ricordato sempre il professor Fiasco, l'interazione tra il gioco legale e quello illegale «si gioca proprio sull'espansione del Il nesso è logico e di intuitiva evidenza, perché è fin troppo ovvio che sono i giocatori compulsivi e patologici le prede più sensibili di questo sistema. Il mancato riconoscimento della patologia e delle possibili conseguenze espone le famiglie di queste persone a lottare, in solitudine, con la criminalità, e a sopportarne i pesanti oneri economici. Lo Stato potrebbe trovarsi in una situazione imbarazzante perché, se dovesse riconoscerla e quindi inserirla nei livelli essenziali di assistenza, dovrebbe proibire ogni forma di pubblicità perché altrimenti si profilerebbero delle responsabilità civili. Ma ancora una volta occorre sciogliere il dubbio amletico di shakespeariana memoria «essere o non essere»: si vuole cambiare rotta oppure si vuole continuare in questo modo? che, se accolta, potrebbe arginare questo fenomeno davvero drammatico: inserire nei livelli essenziali di assistenza le ludopatie. Speriamo che venga fatto al più presto. Lo scopo è quello di garantire la presa in carico delle persone affette da ludopatia che, voglio ricordare, è stata definita dall'Istituto superiore di sanità come una dipendenza senza sostanza, che si caratterizza per la comparsa di vere e proprie crisi di astinenza e con una perdita totale dell'autocontrollo. Come accennavo poc'anzi, la relazione, che è condivisibile sia nel metodo che nei risultati e nelle conclusioni formulate, non tiene in considerazione in modo

perché l'uomo che dovevo sposare è affetto da questa patologia. (...) Dovete denunciare voi stessi, che siete servitori dello Stato, questo sistema di distruzione legalizzata, invece fate i taciti indifferenti. (...) Non credo possa sapere cosa voglia dire dover combattere con un mostro simile, ma mi auguro possa mettersi nei nostri panni. (...)» e poi aggiunge: «con i vizi che ci proponete e ... ci anestetizzate. Non vogliamo rubare, allora finiamo per tentare la fortuna, tanto se non c'è prospettiva, cosa abbiamo da perdere?». È un grido di aiuto, a cui oggi discutendo questa saggia relazione vogliamo rispondere e dobbiamo assumerci la responsabilità di compiere quelle modifiche proposte dalla Commissione,

certamente merita un notevole plauso la relazione che oggi stiamo discutendo, ma, pur nel plauso, assolutamente meritato e indiscutibile, ancorché vi sia una lacuna che poi lacuna che poi espliciterò, mi corre l'obbligo di porre all'attenzione della Presidenza e dei colleghi l'irritualità di questa discussione.

Irritualità nella discussione che porta a un rischio di conflitto tra istituzioni, perché la discussione di una relazione si conclude nell'ambito dell'organismo istituzionale; poi, naturalmente, trattandosi di bicamerale, viene comunicata ai Presidenti di Camera

che ingenererebbe un problema; non in questa occasione, però evidentemente questo è un problema. Allora, questa irritualità nella prassi può portare l'Aula di una delle Camere ad essere ulteriore momento di valutazione dell'attività di una Commissione bicamerale, che invece, torno a dire, deve essere conclusa all'interno di quell'organismo. Questa era la premessa che mi correva l'obbligo di fare. La legge prevede che la Commissione possa proporre dei disegni di legge, che ne prendano atto organismi del Governo e delle Camere affinché si possano incentivare iniziative legislative, promuoverle e renderne più veloce veloce la procedura; ma la valutazione in sé non è possibile. Si può parlare del fenomeno, che è tutt'altra cosa: parliamo del fenomeno del gioco, parliamo del fenomeno delle droghe, tanto per fare un esempio, ma non parliamo della relazione della Commissione antimafia. Ciò posto,

lacuna di cui parlerò tra poco, sulla tematica delle lotterie, dei videogiochi, dei giochi elettronici, dei giochi *on line* e tutto il resto, perché ha affrontato in maniera assolutamente notevole tutta la tematica, evidenziando i problemi complessivi, sia di carattere generale sia di carattere concreto. concreto. Ai giochi la criminalità organizzata è certamente molto interessata, per un motivo semplicissimo: perché è un'attività che non desta allarme sociale ma a cui anzi è molto interessata una certa fascia di società, con tanti cittadini; inoltre non è appariscente come può essere qualsiasi altra attività criminale e dà tantissimo denaro. Quindi è una di quelle attività cui la criminalità organizzata presta particolare attenzione, considerando tra l'altro il gettito che può dare. In un momento in cui c'è un ampio ricorso al gioco, alle lotterie e a tutto il resto per finanziare le casse dello Stato e quindi si ampliano le possibilità di questa attività, evidentemente l'attenzione deve essere particolarmente forte, perché l'attività della criminalità organizzata corre su due binari: quello abituale di carattere estorsivo - l'imposizione ad un gestore di locale pubblico di videogiochi o di altre attività, il prelievo sulle vincite legittime - ovvero quello della falsificazione vera e propria, quando c'è una connivenza col gestore o con il concessionario, dei dati delle vincite, quindi una sottrazione alle casse dello Stato di una parte della vincita.

particolarmente preoccupato perché dà conto di una capacità di attrattiva da parte del mercato illecito di quella che certamente è una debolezza o un ricorso al mercato della speranza.

A fronte di questo, c'è anche un mercato parallelo pericolosissimo di prestiti a tassi usurari, che gioca accanto alla casa da gioco la propria partita. Esso è estremamente pericoloso, in quanto è collegato con vere e proprie sentinelle all'interno della casa da gioco utili ad attrarre lo sfortunato che vuole continuare a tentare la fortuna.

emerge, in ogni caso, un'insufficienza se non una vera propria assenza del sistema dei controlli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sembra quasi che l'Amministrazione recepisca quello che le arriva in maniera assolutamente acritica, senza avvertire la necessità di controllo di quello che accade realmente. E l'esempio fatto dal

Ricorre frequentemente la richiesta di aperture di concessioni a nuovi casinò con la scusa che possono rappresentare momento di attrazione turistica. momento di attrazione turistica deve essere la proliferazione di eventi culturali o l'esaltazione delle bellezze monumentali o paesaggistiche. Questi sono i migliori elementi di attrazione turistica. Non sono certamente i casinò ad attrarre possono soltanto attrarre quel contorno illecito illegale o addirittura esaltare un momento patologico di tanti.

il lotto quotidiano e la possibilità di vincere giocando il giusto, francamente mi lascia molto perplesso. Non mi convince sulla capacità di uno Stato di incentivare altro tipo di attività piuttosto che ricorrere a questo tipo di prelievo da una attività che

il tema in discussione - lo abbiamo sentito dire anche dai colleghi che mi hanno preceduto - è sicuramente importante, molto complesso e soprattutto molto diffuso.

I numeri lo evidenziano. Abbiamo un incremento del ricavato positivo, ma solo da un lato, ossia per le casse dello Stato. Secondo i dati forniti da L'Osservatorio del gioco *on line* del Politecnico di Milano, solo nello scorso anno il fatturato dei giochi *on line* si è chiuso con una crescita della raccolta di oltre il 40 per cento, e credo che questo sia un dato significativo che ci deve

i 1,484 miliardi giocati nel 2009 e i 3,765 miliardi dello scorso anno. gli altri dati, da dicembre scorso ad oggi il numero dei conti di gioco aperti sul *web* da utenti italiani è passato da 2,8 milioni a 4,7 milioni, con una crescita del 70 per cento in soli 7 mesi. Da ciò nasce la forte preoccupazione per questo triste fenomeno, che colpisce molte categorie, soprattutto le fasce più deboli, e in particolar modo i giovani.

il risultato che se ne è ottenuto: un risultato trasversale che ha visto l'impegno e la condivisione di tutti su questo argomento. Ciò sta a significare che, quando la politica si impegna compatta ed unita su un determinato argomento, i risultati alla fine arrivano. Ritornando ai numeri del fenomeno verifichiamo che le entrate derivanti dai giochi si stimano complessivamente sui 7,2 miliardi di euro. Il mercato italiano rappresenta un dato notevole, ossia quasi il 10 per cento del mercato mondiale in quanto a valore e volume di gioco.

In Italia - lo abbiamo detto prima - quelli più coinvolti purtroppo sono i ceti sociali più deboli e meno abbienti, in quanto lo stato di bisogno genera automaticamente una forte e quasi disperata ricerca della fortuna, quale stimola le persone a risolvere i propri problemi economici tentando la strada del gioco. I numeri sono impressionanti: in Italia 2 milioni di persone sono soggette al rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

al contrario, dove il tenore di vita è più alto si gioca di meno: è il caso di città come Biella, Padova, Trieste e altre città del Nord. Il fatturato complessivo del gioco di Stato ammonta a 60 miliardi di euro, pari al 4,5

1,3 ai gestori e 18,7 ai vincitori. Le macchine più diffuse sono le *slot machine,* i *videopoker,* il casinò e i *poker on line:* sono questi i nuovi strumenti della mania del gioco definita tecnicamente, anche dai colleghi, come ludopatia.

sicuramente attendibili della Guardia di finanza, rese pubbliche sulla stampa e avallate dalle testimonianze di vari operatori del settore,

Questa stima viene inoltre correlata al fatto, anch'esso supportato da testimonianze, che nel Paese vi sono oltre 200.000 apparecchi ufficiali

Il problema della dipendenza da videogiochi sta assumendo negli ultimi tempi proporzioni sempre di maggior rilievo, e purtroppo, a seguito di questo, migliaia di persone finiscono sul lastrico per colpa dell'ossessione per le cosiddette macchinette mangiasoldi.

giovani, purtroppo moltissime famiglie del nostro Paese. L'esplosione di questo fenomeno è legata a tanti fattori, primi fra tutti la liberalizzazione del mercato, che sicuramente è uno dei problemi principali, e l'ampliamento delle modalità di gioco, che ha portato al settore nuovi operatori e anche innovazione tecnologica.

incidenza tra le ragazze. Gratta e Vinci, lotterie istantanee, scommesse sportive, Lotto e Superenalotto sono i giochi che vengono maggiormente praticati. I minorenni scolarizzati che scommettono illegalmente sono più di mezzo milione, una cifra veramente impressionante. L'aumentare del fenomeno ha naturalmente fatto emergere una versione più evoluta dei cravattari, cioè coloro che prestano denaro a strozzo. Accade quindi che i cosiddetti prestiti già da qualche tempo siano concessi per finanziare le giocate, fenomeno che coinvolge direttamente sia gli operatori economici, sia i commercianti che anche, a volte, i piccoli imprenditori.

Va senza dubbio posto un freno a questa situazione, allo smodato utilizzo del gioco d'azzardo e del *videopoker*, anche perché il gioco d'azzardo alimenta altri circuiti criminali come l'usura e il riciclaggio.

Si impone pertanto una riformulazione o comunque un'integrazione all'articolo 88 del Testo unico attualmente vigente che tenga conto delle pronunce interpretative della Corte di giustizia europea, fatte proprie dalla Corte di cassazione. Ben venga quindi il lavoro svolto in Commissione antimafia e ben vengano anche le proposte avanzate dalla Lega Nord, che ha contribuito a pieno titolo a questa risoluzione.

consapevolmente immaginabile che questa persona potesse risiedere in un territorio già fortemente compromesso da altri recenti provvedimenti

Grazie al lavoro di tutti, questa persona, ritenuta dai più indesiderata, è tornata a casa sua.

la lettura di questo documento genera un senso di soddisfazione parlamentare. Scopro, come lettore, che un'attività ben indirizzata può produrre un approfondimento conoscitivo di cui all'inizio ignoravo lo spessore. Si vengono a sapere tantissime informazioni, ma soprattutto c'è anche un quadro conoscitivo organizzato che permette anche la continuazione di uno studio ulteriore. Se posso fare un paragone forse un po' strano, leggendo questa relazione mi è venuta in mente l'inchiesta agraria di che in anni lontanissimi ha dimostrato che quando l'attività parlamentare è rivolta all'approfondimento della conoscenza di un tema può dare contributi preziosi, che restano non solo negli annali del Parlamento ma anche nella cultura collettiva della società. La relazione ci illumina sulla connessione strettissima tra il gioco legale e quello illegale: è difficilissimo trarre una linea di demarcazione. Il gioco illegale chiama in causa le multiformi presenze della criminalità organizzata, e questo determina un avvitamento particolarmente preoccupante. In realtà, però, la relazione ci fa vedere con occhio severo anche semplicemente la dimensione del gioco legale.

in numerosi loro interventi, anche se non fosse distorto e mistificato dall'azione dell'attività illegale, sarebbe già di per sé un argomento su cui approfondire la conoscenza e prendere le misure Questa relazione fa capire anche a chi non sa nulla che è il 1992 l'anno in cui lo Stato cambia stile. Prima del 1992, il gioco era sostanzialmente confinato all'interno all'interno di ambiti particolarmente ristretti, quasi elitari. E la natura censurabile del gioco d'azzardo era in un certo senso illuminata e confinata all'interno Le esigenze dell'erario dal 1992 in poi hanno incrementato vistosamente una dilatazione sempre più incontrollata delle occasioni da gioco con uno schema ben fotografato da uno dei testimoni delle associazioni antiusura quando parla di una chiara imposta regressiva sul reddito.

incrementa vieppiù questo tipo di dimensione. Questo rappresenta un'imposta regressiva sul reddito perché si colpiscono proprio i titolari di redditi bassi o nulli, con

con grande efficacia la differenza tra il gioco del povero e quello del ricco, del possidente che deve dimostrare di non voler vincere: il ricco gioca per puro *divertissement* e non deve dimostrare di essere attaccato alla vincita, anzi, quando vince deve ostentare il disprezzo per la vincita; il povero, il il povero, il plebeo che gioca in luoghi sordidi, repellenti, con compagnie discutibili è invece vistosamente attaccato all'elemento della vincita,

i plebei giocano dappertutto, guadagnano pochissimo e impegnano il poco che guadagnano. Su questo punto faccio una connessione arbitraria, passando da Dostoevskij alla tabaccaia da cui vado a comprare il "veleno" dei miei sigari toscani, che è un ottimo sensore sociologico. Se al posto di vendita del tabacco c'è una persona consapevole e ricca di umanità e di sensibilità, quella è un sensore sociologico fondamentale. È qualche anno che, quando vado a comprare i tabacchi da questa signora, ricevo costantemente, tutte le volte, una sorta di fulminea fotografia del dilagare incontrollabile dello spreco dei bassi redditi.

coincide con il giorno della riscossione delle pensioni; egli sarà contento di sapere che il mio sensore sociologico, prima ancora che lui me lo dicesse, aveva già espresso con precisione questo concetto. Addirittura c'è chi si fa dare prestiti da parenti o fidanzati per per accedere al gioco, magari, con due giorni d'anticipo rispetto al momento in cui riceve lo stipendio o la pensione. Nel mio

l'unanimità, così esaltata da tutti che quelli che hanno parlato, ha un senso, e se davvero tutti nella Commissione sono stati concordi nel prendere l'impegno solenne di intervenire nelle forme che sono state dette (modifica della legge e progetti di disegni di legge più incisivi sull'argomento), il problema non è se si sottopone al voto o no una relazione, e si può arrivare a smentire con l'Aula l'operato della Commissione bicamerale, ma è molto più semplice. Se davvero la Commissione bicamerale ha espresso un punto di vista unitario e forte su questo punto, questo si traduca semplicemente nell'azione consapevole delle Aule parlamentari nell'approvare con la massima rapidità e con la massima decisione le modifiche che sono state proposte. Non c'è trucco, e, anzi, dirò di più: tutti i membri della maggioranza, che hanno sentito con passione questo argomento, s'impegnino a bocciare le eventuali iniziative del loro Governo, nel caso in cui esso È molto semplice, cari colleghi; siete d'accordo? Agite di conseguenza. L'irritualità è formale, ma l'elemento fondamentale è la volontà sostanziale. Tale volontà, per esempio, non può arrivare arrivare ad accettare il solletichío dilettantesco del Presidente del Consiglio che, sbarcato a Lampedusa, altro non sa dire che si comprerà la villa e, quasi quasi, ci farà anche una casa da gioco.

censurata con una risata, ma anche contraddetta da una pratica comune e seria di entrambe le Assemblee legislative.

dati, signora Presidente e colleghi senatori,

La circostanza che noi si sia qui oggi e che il Gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere, insieme agli altri Gruppi, abbia chiesto la calendarizzazione di questa relazione, facendo proprie una serie di iniziative parlamentari, a cominciare da quella *bipartisan* che vede come primo firmatario il senatore Lauro e tanti altri colleghi di maggioranza e opposizione, non è un rito, non è un'innovazione rispetto a una prassi parlamentare: si tratta dell'esigenza di mettere al centro della discussione parlamentare una questione estremamente grave e di importante attualità per il nostro Paese. Come dirò, mi auguro brevemente, nel corso del mio intervento, ci troviamo di fronte alla circostanza che affidiamo al gioco una parte consistente delle entrate del bilancio dello Stato, e per fare questo tolleriamo fenomeni di illegalità diffusa che stanno attorno a questa situazione e che devono essere oggetto di una regolamentazione. se pensiamo che comunque il Parlamento e le istituzioni hanno anche una funzione, non voglio dire educativa, perché mi sembra fin troppo impegnativo, ma che comunque può incidere su usi e costumi della nostra comunità, che ci fanno sempre più diventare, lo dico in maniera assolutamente convinta, più simili ai Paesi dell'ex Unione Sovietica in cui l'alcool e il gioco sono gli unici strumenti di coesione sociale. Credo che su questo tema bisogna tutti fare meno dispute di carattere regolamentare e formale e invece renderci conto che in questo momento, anche e soprattutto di crisi della nostra economia,

del fenomeno del gioco d'azzardo, con particolare riferimento a quello lecito e a quello illecito, e ha approvato all'unanimità due relazioni

specifica il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito. In queste relazioni è chiaramente evidenziato un catalogo di criticità del sistema, in quanto il gioco d'azzardo costituisce il punto di incontro di gravi distorsioni dell'assetto socioeconomico socioeconomico del nostro Paese: l'esposizione dei redditi degli italiani al rischio dell'erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione all'arricchimento ad ogni costo di taluni concessionari che operano in regime di oligopolio; il collegamento diretto con fenomeni criminali quali l'usura, l'estorsione, il riciclaggio; la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Soprattutto, emerge come nei periodi di crisi economica come quello che stiamo drammaticamente vivendo il gioco di azzardo sia utilizzato come strumento di imposizione indiretta e mascherata. Non potendo infatti forzare i limiti fisiologici dell'imposizione fiscale, il Governo e l'erario favoriscono il ricorso all'incentivazione della malattia del gioco, con un meccanismo che favorisce «forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento»: così, testualmente, dice la relazione (dobbiamo cominciare anche a mettere un po', come si suol dire, i piedi nel piatto). Non si comprende bene il quadro che abbiamo davanti se non si ricordano i dati del settore, come peraltro riferiti nelle varie relazioni della Commissione antimafia. La raccolta dei giochi in Italia tra il 2003 e il 2010 è stata complessivamente di 309 miliardi di euro e il comparto dei giochi pubblici e delle scommesse sportive è diventato il settore trainante delle finanze del Paese. I volumi di raccolta delle scommesse sono aumentati ad un tasso medio annuo del 23 per cento tra il 2003 e il 2009, passando da 15,4 a 54,3 miliardi di euro, e del 13 per cento nel 2010, raggiungendo la cifra di oltre 61 miliardi di euro, cioè più del 296 per cento rispetto al 2003, con una proiezione per il 2011 di oltre 70 miliardi di euro. Le corrispondenti entrate erariali sono state pari a 8,733 miliardi di euro, ma sono diminuite rispetto all'anno precedente di circa lo 0,8 per cento, a fronte di un incremento della raccolta pari al 13 per cento, con la previsione di un incremento dello 0,2 per cento per il 2011: sembra quasi che le entrate in ribasso denotino una sorta di pudore dello Stato che potremmo definire, così come fa la Commissione, «biscazziere». Sì, uno Stato biscazziere, perché si mostra interessato solo alle entrate e disinteressato rispetto alle questioni sociali e di illegalità connesse al gioco d'azzardo. Dobbiamo con forza sottolineare che l'aumento del fenomeno del gioco patologico tra i giovani sembra essere considerato un problema di interesse pubblico solo all'estero, ma non in Italia. ha ben sottolineato la relazione oggi al nostro esame: «in concomitanza con il proliferare dei giochi d'azzardo, anche *on line* ed a bassa soglia d'accesso, in tutto il mondo si sta sviluppando l'interesse degli studiosi circa i costi sociali, economici e psicologici, associati al gioco eccessivo, specie nei giovani; le attuali norme vigenti ed i sistemi di controllo, in Italia, non garantiscono concretamente la tutela dei minori» - come non la garantiscono nel settore dell'uso e dell'accesso alle sostanze alcoliche e superalcoliche «che accedono liberamente a luoghi loro vietati, a causa della irrisorietà delle sanzioni a carico degli esercenti infedeli; intorno ai luoghi del gioco d'azzardo, anche lecito o autorizzato, nei quali accedono spesso liberamente i minori, si creano circuiti criminali, collegati all'usura, al riciclaggio del danaro sporco e allo spaccio degli stupefacenti; non esistono protocolli sanitari, né strutture idonee al recupero di giocatori patologici, specie giovani».

Le ludopatie, il gioco d'azzardo compulsivo, che colpiscono molto più spesso le fasce deboli e meno abbienti della popolazione con un effetto moltiplicatore dei danni economici e sociali della patologia da gioco, hanno risvolti sociali tragici.

«Le cause che generano l'usura dovrebbero essere tutte prevenute e non incentivate, come invece accade ad esempio con il gioco d'azzardo. (...) Anche la questione dei giochi per l'Abruzzo mi pare significhi salvarsi in *corner*. Ogni volta che c'è bisogno di fondi, si ricorre al gioco d'azzardo e questo mi sembra anche immorale. Non lo dico perché sono un prete (ma gioisco dell'esserlo), lo affermo soprattutto come uomo: è un principio sballato, che non tiene affatto in conto gli studi svolti da sociologi e psicologi sull'argomento. Non vorrei che capitasse quello che è accaduto per il fumo: adesso sui pacchetti di sigarette si scrive che il fumo uccide perché i soldi non sono più sufficienti per curare le vittime del fumo. Presto, anche i soldi incassati con il gioco d'azzardo non saranno più sufficienti per curare le vittime del gioco d'azzardo. Attualmente, a fronte di una popolazione dell'80 per cento di italiani che giocano, i giocatori patologici costituiscono oltre il 3 eppure l'incremento di tale percentuale si facilita in tutte le maniere, non so con quale senso di moralità e di servizio alle persone». L'analisi della normativa di controllo e di contrasto agli abusi ed alle illegalità ha mostrato ampie ed irrisolte falle. Si pensi alle inefficienze dei sistemi di controllo. Il professor Fiasco, consulente della Consulta antiusura, ha riferito che quasi ad ogni operazione di controllo sui gestori ed operatori del settore corrispondeva un risultato positivo, nel senso dell'accertamento di un caso di abuso (in particolare, di disconnessione delle macchine per il gioco dal sistema centrale di controllo della SOGEI), ma ha riportato anche dati numerici intollerabili: a Roma ci sarebbero sei addetti che si occupano dei controlli in tutta la Polizia di Stato, quasi altrettanti nella Guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri e quasi nessuno nella Polizia municipale; in totale, vi sarebbero solo 20-30 persone addette ai controlli, a fronte di 70.000-80.000 postazioni dislocate su un enorme territorio. I costi sociali del fenomeno possono essere valutati nel loro complesso solo in una visione integrata dell'impatto e delle ricadute del gioco, e sono rappresentati da diversi risultati indotti: il primo è la redistribuzione della domanda di beni e servizi; il secondo è l'incentivo alla criminalità comune e organizzata; il terzo è il dirottamento delle risorse finanziarie locali, poiché l'allocazione del risparmio per finalità produttive viene convertita in attività parallele (e non di rado illegali) al gioco d'azzardo. Dal punto di vista dell'illegalità diretta, il rischio maggiore è rappresentato dall'uso del gioco d'azzardo per il riciclaggio di capitali sporchi. E tale pericolo è tanto maggiore nel nostro Paese quanto più è strutturata la presenza di organizzazioni di tipo mafioso. Signor Presidente, sin dalla loro costituzione, gli organismi internazionali di azione contro il riciclaggio hanno indicato il pericolo rappresentato dal ricorso ad «intermediari finanziari non tradizionali», da parte della criminalità organizzata. force*) valuta che occasioni privilegiate per le operazioni di occultamento dell'origine della ricchezza si trovino tra i casinò, nelle lotterie, nelle sale da gioco, tra gli uffici di cambio e tra gli uffici di trasferimento fondi, nei servizi per l'incasso di assegni, nei corrieri e tra i grossisti di gioielli e di pietre preziose e tra i venditori di opere d'arte: tutti soggetti che forniscono servizi finanziari di tipo bancario, pur essendo sottoposti a regolamentazioni e controlli assai più limitati rispetto ai tradizionali operatori finanziari. In Italia, il sistema appare poi particolarmente permeabile ad interventi della criminalità organizzata, anche per carenze strutturali ed organizzative che incidono sulla complessiva efficienza del sistema pubblico di riscossione dei diritti erariali e sui controlli di legalità. Appare evidente come l'attuale normativa in materia sia finalizzata ad applicare le norme antiriciclaggio alla quasi totalità dei giochi d'azzardo legali, ma è altrettanto evidente che nel settore dei controlli si sconta il rischio maggiore della violazione delle regole: prevedere regole di identificazione del giocatore

dei controlli si sconta il rischio maggiore della violazione delle regole: prevedere regole di identificazione del giocatore o di segnalazione di operazioni sospette a carico del gestore senza poi sottoporre le procedure di gioco legale a controlli periodici ed i contravventori alle regole a sanzioni severe significa, di fatto, non creare alcuna sostanziale barriera al riciclaggio. Allo stesso modo, appare sempre maggiore negli anni l'interesse della criminalità organizzata al settore del gioco (in particolare quello lecito), proprio per utilizzarlo come strumento di riciclaggio e lavaggio di denaro sporco. Il gioco d'azzardo è attività tradizionale delle associazioni mafiose, in passato molto impegnate nella diretta gestione delle bische clandestine ricordare l'estensione del fenomeno a Milano negli anni 1960-1980) e poi in altri esperimenti di imprenditoria illegale collegati alle scommesse (ad esempio, il cosiddetto Totonero, ossia la riedizione in salsa mafiosa del Totocalcio). Secondo la Direzione nazionale antimafia «la criminalità non si è lasciata sfuggire l'occasione di insinuarsi anche in attività relativamente recenti, come la gestione delle sale Bingo. Le scommesse clandestine e le sale Bingo continuano a rappresentare settori di interesse per la criminalità organizzata, sia per quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di gestione delle sale Bingo, che si prestano costituzionalmente ad essere un facile veicolo di infiltrazioni malavitose e di riciclaggio, sia per quanto riguarda le società concessionarie della gestione della rete telematica, dove si è assistito ad un duplice fenomeno: da un lato l'aggiudicazione a prezzi non economici di talune concessioni e, dall'altro, al proliferare dei punti di scommessa, i cosiddetti *corner*, alcuni dei quali chiaramente inseriti in una rete territoriale dominata dalla presenza di un circuito criminale Il fenomeno rischia di assumere ora una portata assai più rilevante, tanto per ciò che attiene alla distribuzione territoriale, quanto per ciò che riguarda i valori economici dell'investimento mafioso. Ciò per un duplice ordine di fattori: da un lato, la legalizzazione del gioco d'azzardo con le *slot machine* (sancita dalla 1egge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria del 2003) ha allargato enormemente ed esteso ad ogni angolo del territorio nazionale il bacino d'utenza; d'altro canto, l'enorme crescita economica di alcune lotterie, come il Superenalotto, ha reso appetibili per le organizzazioni criminali tali sistemi per finalità di comodo riciclaggio. Oggi, come sottolinea una recente analisi della Direzione nazionale antimafia «il gioco, per i notevoli introiti che assicura a fronte di rischi "giudiziari" relativamente contenuti, è ormai diventato la nuova frontiera della criminalità organizzata di stampo mafioso». Ciò anche per le dimensioni economiche complessive del fenomeno, che nel nostro Paese hanno assunto caratteri numericamente e percentualmente rilevanti. La relazione ricorda che «l'Italia è tra i primi cinque Paesi al mondo per volume di gioco: l'industria del gioco ha attualmente un fatturato complessivo pari al 3 per cento del PIL e dà lavoro a 5.000 aziende e 120.000 persone. Tali dati, che si riferiscono al gioco legale, sono destinati ad impennarsi se si guarda anche al gioco clandestino». Il meccanismo illecito che si riscontra in maniera diffusa consiste, pertanto, nell'alterare i flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco dalle macchinette al sistema di elaborazione del concessionario, ovvero ad intervenire direttamente sui contatori per ridimensionare l'entità dei dati di gioco. In tal modo la criminalità si appropria sia degli importi che dovrebbero essere corrisposti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta, sia dell'aggio del concessionario, che è ovviamente proporzionale al volume delle giocate. Questo sistema si fonda su enormi, macroscopici ed ingiustificati difetti nei sistemi di controllo, peraltro nemmeno di recente datazione. Basterebbe citare, ad esempio, come fanno le relazioni della Commissione antimafia, gli esiti della cosiddetta Commissione Grandi del 2007, ossia della «Commissione d'indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento, e per l'analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi» istituita dal Ministero dell'economia durante la XV legislatura e presieduta dal sottosegretario Grandi. Quella Commissione verificò che nel corso degli anni precedenti erano state commesse dai concessionari dei servizi plurime violazioni delle regole, con mancato versamento dei diritti erariali per svariate centinaia di milioni di euro. Inoltre, sulla base dei dati oggettivi e delle valutazioni della Guardia di finanza, essa stimò che nel corso degli anni 2003-2006 il numero delle *slot machine* abusive - ossia operanti pur non connesse al sistema informatico di controllo - andasse dalle 100.000 alle oltre 200.000. Infine segnalava che diverse fonti rendevano «evidente l'interesse della criminalità organizzata verso questo settore, che è quindi soggetto a rischi di infiltrazione La stessa relazione segnalava ancora un dato numerico inquietante: nell'anno 2006, a fronte di una raccolta del gioco lecito pari a 15 miliardi e 400 milioni di euro, la raccolta del gioco illecito sarebbe valutabile in circa 43 miliardi e mezzo di euro (stima della Guardia di finanza). A fronte di questi dati, a fronte anche delle iniziative della Corte dei conti, che ha avviato un'azione di responsabilità di responsabilità - in concomitanza dei lavori della commissione Grandi - nei confronti delle società concessionarie, con contestazioni di addebito di responsabilità superiori a 90 miliardi di euro (tra somme dovute, sanzioni ed interessi), una cifra francamente sbalorditiva e che rende l'idea dell'enormità del fenomeno, ci saremmo aspettati, al di là del dibattito e della relazione, un intervento da parte del Governo e della maggioranza su questo tema.

questo tema coinvolge questioni di natura economica, ma soprattutto questioni di natura sociale che sono aperte, rispetto alle quali noi assistiamo impotenti all'atteggiamento cinico di chi dice «*pecunia non olet*»: purché si tratti di soldi e purché con questi manteniamo il bilancio dello Stato, non ci dobbiamo porre il problema di come questi soldi vengono riscossi, a quanto ammontano e chi illegalmente sfrutta i giovani con questi metodi.

che contrastano il gioco d'azzardo, a partire da quella presentata dal collega Lauro, che il Gruppo parlamentare da me presieduto ha fatto propria e di cui ha chiesto l'inserimento in calendario. Questo dibattito, infatti, non è un rito inutile: questo dibattito serve se è funzionale ad aprire in Parlamento una discussione sulle proposte di legge e a fare in modo che il Parlamento intervenga, malgrado il cinismo e l'assenza del Governo su questa materia.

segmento giochi: «Il gioco, per i numerosi introiti che assicura, a fronte dei rischi giudiziari relativamente contenuti, è diventata la nuova frontiera della criminalità organizzata di stampo mafioso».

come hanno correttamente sottolineato sia il coordinatore del VI Comitato Li Gotti che il collega D'Alia, un tema che investe ormai una parte rilevante del nostro Paese. Credo, che venga ampiamente sottovalutato che cosa è oggi il gioco d'azzardo lecito nel nostro Paese. Alcuni macrodati sono stati già forniti e sia

Sono stati forniti dati complessivi, ma se li guardiamo nel *trend* di sviluppo decennale, essi sono forse anche più significativi. In dieci anni la spesa per consumo di gioco nel nostro Paese è passata da 6 a 60 miliardi. Io credo che nessun altro genere

cento dell'ammontare complessivo della spesa per consumi degli italiani è destinato al gioco d'azzardo lecito, per tralasciare poi quello illecito, su cui tornerò successivamente.

In 20 Province italiane, adeguatamente sparse su tutto il territorio, la percentuale di PIL *pro capite* impiegata nel gioco d'azzardo è superiore al 5

gli investimenti pubblicitari fatti dai vari soggetti che operano nel settore per indurre ad incrementare la partecipazione al gioco d'azzardo lecito sono considerevoli. Sia dalla Sisal che da Lottomatica sono stati forniti dati in ordine di svariati miliardi investiti

Le entrate erariali che sono conseguite a questo nuovo approccio al gioco da parte dello Stato nell'ultimo anno sono state ai 9 miliardi di euro, contro i 3,7 miliardi di euro del 2001. Credo che nessun'altra entrata dello Stato abbia avuto un incremento di questa natura. È un fenomeno che, nella sua espansione, ha Grazie, più o meno 1.600 aziende, con un fatturato medio di oltre 4 milioni di euro e un valore aggiunto di 1,5 milioni di euro, che si occupano Sto parlando di coloro che costruiscono macchine da gioco, di coloro che producono i Gratta e Vinci: quindi di tutto l'indotto che ruota intorno all'azienda Non va sottovalutato poi che queste aziende investono in ricerca e sviluppo più o meno lo 0,6 per cento del fatturato, che è quasi il doppio della media degli investimenti degli altri settori. che dà lavoro a 14.000 addetti, senza contare i 70.000-80.000 delle reti tradizionali delle ricevitorie che, da sempre, operano nel settore. Per concludere su questo punto, il quadro che è emerso dalle indagini che abbiamo svolto all'interno del Comitato ci dà un Paese in cui 35 milioni di persone giocano almeno una volta l'anno, a testimonianza di un livello di diffusione amplissimo, con una raccolta che si attesta nel 2010 (sono gli ultimi dati certificati che abbiamo) intorno all'11 per cento del PIL, con il risultato che l'industria del gioco è la terza industria italiana dopo l'ENI e la FIAT.

legale/illegale nell'ambito del gioco d'azzardo. L'assunto secondo il quale l'incremento del gioco d'azzardo lecito avrebbe nel Grazie,

con modalità del tutto nuove. Aspetto, questo, estremamente interessante e da approfondire, anche alla luce delle modifiche normative da approntare. Le nuove modalità di gioco hanno

il gioco pubblico d'azzardo è diventato una grande leva per fare cassa, con il 32 per cento sul consumato. Come ha significato il collega Li Gotti prima,

l'introduzione dei nuovi giochi e quindi consolidare il gioco d'azzardo lecito su tutto il territorio nazionale, si è provveduto a una sorta di alleggerimento fiscale, che comunque assicura sempre un considerevole introito Credo proprio che oggi si possa dire che il gioco è un'entrata di cui questo Paese, essendosi strutturato in questa direzione, non può più fare a meno. In sostanza, i nostri saldi di bilancio sono ludodipendenti. Si tratta di un'entrata certa, che aumenta considerevolmente di anno in anno. Non sottovalutiamo però a questo riguardo che comunque si tratta di 60 miliardi di euro sottratti ad altri consumi. E non è neanche detto che lasciati ad altri consumi porterebbero minori entrate per l'erario, perché, se consideriamo che più o meno cento di questi consumi torna o resta nell'erario dello Stato, lasciato ai consumi ordinari a cui viene sottratto probabilmente porterebbe, tra oneri sociali, imposte dirette e indirette, maggiori entrate per il circa 30 per cento: così è stato stimato. Inoltre, veniamo già state sottolineate da molti senatori che mi hanno preceduto le problematiche sociali che si collegano al gioco d'azzardo lecito. Non va sottovalutato e su questo credo che tutti abbiano cercato di richiamare l'attenzione dell'Aula e mi auguro con successo - che oggi stiamo parlando di un fenomeno che rischiamo di leggere con occhiali vecchi. Infatti il gioco c'è sempre stato (è dal 1200 che lo Stato è biscazziere, da quando ha scoperto che potendo regolamentare il gioco diventava un giocatore che faceva le regole),

il fenomeno del gioco lecito gestito dallo Stato. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Intanto, se per circa cent'anni lo Stato biscazziere si è comportato nello stesso modo, comunque avendo prudenza e considerando

dagli anni Novanta in poi c'è stata una caduta di questa riserva etica nei confronti del gioco. Questo ha aperto nuovi orizzonti negativi, che hanno come collaterale tutta la patologia del gioco, dall'usura alle appropriazioni indebite alle assenze dal lavoro a tutti quei fenomeni che sono stati anche in parte ricordati oggi che sono generalmente etichettati come fenomeni di ludopatia e quindi di devianza. senza sottovalutare il fatto della rilevanza del rapporto intergenerazionale. Una recente ricerca di Nomisma, che ha un osservatorio su questi fenomeni ci dice che,

dobbiamo attrezzarci ad avere un approccio diverso nella lettura del gioco lecito. Diverso perché sono

se si possa utilizzare questa sensibilità tutta italiana riconosciutaci al gioco e trasformarla in uno strumento di lotta all'evasione fiscale, aumentando la *tax possibile che il gettito fiscale potrebbe aumentare se i tradizionali scontrini fiscali fossero sostituiti da ricevute attestanti la partecipazione a concorsi o lotterie? La Cina lo sta sperimentando con risultati estremamente positivi.

Centaro - questa discussione. Parlare di irritualità di fronte a un tema così drammatico, che investe il futuro stesso del nostro Paese, mi è parso veramente stupefacente. Come stupefacente mi è parso il rilievo sulla lacuna della relazione. Nella relazione saranno contenute altre lacune, ma la lacuna in Non c'è perché, nelle proposte legislative in essa contenute (vero, senatore Li Gotti?), ci sono le proposte del tracciamento di tutte le scommesse, del registro delle scommesse e dell'individuazione di quali società sono alle spalle dei concessionari. Quindi, vorrei partire dalla coda. Chiedo al presidente Schifani e alla Conferenza dei Capigruppo, come ha già anticipato il senatore D'Alia, che ringrazio personalmente (e non perché il gioco sia un problema mio: il gioco è un problema nazionale, non del senatore Lauro!), che venga calendarizzato al più presto possibile l'insieme dei disegni di legge presentati da senatori della maggioranza e dell'opposizione riguardanti le misure urgenti per la tutela dei minori, per il divieto di pubblicità ingannevole, per il tracciamento delle scommesse e per le norme antiriciclaggio. Ma queste misure urgenti sono solo una fase. Ce n'è un'altra, e più importante, sulla quale in quest'Aula si pronunciò anche il Governo tramite il sottosegretario Giorgetti: quella cioè di una riforma organica del settore del gioco, che affronti tutti gli aspetti, e che non può più attendere. Infatti, le nostre norme sono assolutamente inadeguate e insufficienti, e la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può, con le norme attuali, combattere l'infiltrazione mafiosa, che c'è nel gioco illecito ma c'è anche nel gioco lecito, perché sui territori criminali la sovranità criminale controlla attraverso dei prestanomi quasi tutte le agenzie di scommesse. Occorre una riforma organica che affronti tutte le componenti del sistema: quelle amministrative, quelle economiche, quelle di pubblica sicurezza, quelle di controllo di gestione dei mercati finanziari,

quali sono i rischi importati dal comparto dei giochi*on line* attraverso il conto di gioco, quello che nelle nostre proposte, relatore il senatore Li Gotti, viene controllato attraverso i conti dedicati?

attengono agli ambiti: a) strategico e di *governance*, in quanto la presenza dei fondi di *private equity* nell'azionariato dei concessionari può rendere più incerti gli assetti di governo e indirizza le linee strategiche alla massimizzazione del profitto anche attraverso politiche commerciali aggressive;

il problema è che il mercato, come hanno dimostrato tutti i validi interventi fin qui fatti, si è esteso a dismisura, da 10 a 73 miliardi a fine 2011. norme amministrative di controllo non bastano più, né possiamo imputare la responsabilità ai Monopoli di Stato se non esistono norme cogenti e adeguate, né se vi è un sistema di controllo che, sottratto alle forze di polizia e affidato ad ispezioni, si presta, sul territorio, a condizionamenti corruttivi e ricatti personali e familiari da parte della criminalità organizzata. Io invito i miei colleghi senatori, che ringrazio per la loro presenza, ad andare in una delle sale da gioco presenti sul territorio nazionale, nelle periferie delle città, nel Mezzogiorno o in un bar, dovunque ci siano delle postazioni da gioco. All'esterno, dopo le denunce dell'Antimafia, compare un avviso: «Vietato ai minori»; all'interno, tutti quelli che giocano sulle *slot machines* A Las Vegas, il regno del gioco mondiale, se la polizia entra in una sala giochi

Se osservate bene, inoltre, fuori dalle sale da gioco non troverete solo gli usurai che hanno il paccotto da 10.000 euro in tasca per finanziare anziani e meno anziani nel gioco ma anche gli spacciatori di droga, che osservano attentamente i giovani applicati al gioco e li utilizzano organicamente per la consegna delle dosi di cocaina a domicilio; utilizzano questi giovani, finanziati *ad horas*, per le consegne. Quindi, non c'è, cari colleghi, solo il circuito

vedete una persona anziana, uomo o donna, che gioca compulsivamente per delle ore vi accorgerete che, dopo un certo

danni. Ho citato questi esempi perché qualcuno superficialmente pensa che il nostro Paese possa diventare una grande Las Vegas.

ciò significherebbe che la peste del gioco d'azzardo contribuirà a gettare il nostro Paese in un baratro senza ritorno.

Qual è la presenza di gruppi italiani e stranieri e quante le compartecipazioni, o le totali proprietà, di società investitrici registrate in Paesi o città Stato *off shore*? È possibile che i Monopoli di Stato non siano ancora in condizione, con la norma prevista a conclusione della relazione, di sapere chi c'è dietro queste società, che diventano concessionarie e monopoliste e che fanno una pratica della pubblicità anche sulle reti televisive che tutti voi conoscete, quando non si sia passati già agli adescamenti *on line*?

Ci sono alcune società del gioco *on line* che offrono via *e-mail* un accredito di cinquecento, mille euro, un adescamento vero e proprio ad entrare nel sistema del gioco e a non uscirne più.

Paradossalmente in questi anni, di fronte all'espansione del mercato, vi è stato un ridimensionamento delle procedure tradizionali, con grave sottrazione di potere e di controllo all'autorità di pubblica sicurezza. Il senatore Li Gotti ha proposto in calce alla relazione la modifica di un articolo del Testo perchè rimetterebbe in moto anche quei controlli a monte e non a valle, e quindi anche in funzione antimafia, e l'attribuzione di funzioni ispettive, come ho accennato prima, ad entità facilmente condizionabili, specie sul territorio, da pressioni della criminalità organizzata. Questi controlli sono esposti alla pressione di minacce fisiche e di offerte di corruzione. Dobbiamo capire che sono in gioco miliardi di euro e che la pressione corruttiva di questo danaro dilaga senza possibilità di controllo, o per minacce o per offerte corruttive, come dimostrano tutte le indagini della magistratura. Quale argine può essere dato ad un corpo ispettivo, anche se limitato nel numero e nelle entità? Ai concessionari ed ai gestori del gioco pubblico d'azzardo è stato poi aperto il campo alla promozione, all'istallazione capillare con modalità di gioco pubblico d'azzardo, nell'assenza totale di un profilo di responsabilità verso i clienti che invece, come ho detto prima, negli Stati Uniti figura del gestore, del concessionario, dell'intermediario, del responsabile del soggetto affetto da gioco patologico. Se non lo distoglie, non lo allontana, non lo salvaguarda, è responsabile sul piano penale, ma ancor più sul piano civile. La famiglia chiede risarcimenti, talvolta milionari, alle sale da gioco. Sui benefici dell'erario è già stato detto. È chiaro che in una fase di crisi economica come quella che viviamo, se oggi la spesa *pro capite* per ogni italiano euro 1.200, è ipotizzabile che, in una fase recessiva e depressiva del sistema economico

spendere 1.200 euro l'anno per il gioco. Allora tutto il sistema, come accade per la domanda aggregata in momenti di crisi economica, crollerà, e crollando la domanda aggregata di gioco per questa compressione dei redditi, per il processo di indebitamento che c'è stato anche nelle famiglie giocatrici, è chiaro che crollerà

delle entrate e al conto da pagare rispetto ai costi sociali di questo fenomeno.

però importante - e voglio dirlo al senatore Centaro - che ci si trovi allineati nei riti e nelle prassi parlamentari. La Commissione bicamerale antimafia ha presentato in calce delle proposte legislative che, a questo punto, devono essere assegnate, calendarizzate discusse con misure urgenti sui punti che ho richiamato, perché, se non possiamo tornare indietro, almeno rinnoviamo con misure urgenti la tutela dei minori, delle categorie deboli, il divieto di pubblicità ingannevole, il controllo del riciclaggio del danaro sporco, con il registro delle scommesse e con i conti dedicati.

ai responsabili amministrativi dei Monopoli di Stato il compito di emanare decreti per dilatare ancora di più il mercato del gioco. Ho sostenuto la tesi che quella norma

osservazione amara, a fronte di quello che andava discutendo ed approvando la Commissione antimafia,

alla sua intelligenza politica e alla sua sensibilità democratica, e alla Conferenza dei Capigruppo di assegnare urgentemente questi disegni di legge, richiamati dal senatore D'Alia, il cui esame non può più attendere. finestra"). Onorevoli colleghi, il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale è convocato per le ore 15. Qualora non venisse raggiunto il *quorum*, il Parlamento in seduta comune sarà riconvocato alle ore 18,30. Di conseguenza, la seduta pomeridiana del Senato avrà inizio alle ore 16 anziché alle ore 16,30. tribune una delegazione dell'Istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. A loro va il saluto dell'Aula.

nel senso che tutti gli interventi hanno arricchito la relazione su cui ho intrattenuto l'Aula all'inizio di seduta. *(Applausi

Signor Presidente, solo alcune considerazioni per manifestare anche la presenza del Governo a questo dibattito, così interessante, approfondito e ricco di spunti e di occasioni di dialogo e confronto istituzionale.

a quelle norme che il senatore Li Gotti ha indicato in allegato e che dovrebbero portare ad una revisione del meccanismo amministrativo e gestionale di questo settore, legato ai controlli e alle norme. È indubbio che l'attività di gioco è cambiata; forse eravamo abituati nei nostri ricordi di infanzia ad avere quattro case da gioco alle quali pochissime persone potevano accedere, dovendosi comunque spostare; eravamo abituati alla lotteria nazionale legata alle canzoni e forse a qualche lotteria intercomunale o interparrocchiale. Oggi il fenomeno si è destrutturato, quindi l'offerta è molto ampia, molto più grande e ci coinvolge probabilmente

Grazie,

oltre 8.000, con un incremento anche rispetto all'anno precedente, i soggetti verbalizzati; sequestri per strumenti di videogioco, punti di raccolta scommesse, somme in denaro immediatamente recuperate.

hanno portato alla costituzione di una vera e propria polizia dei giochi e delle scommesse. Gli interventi sono tanti e riguardano tutte le parti d'Italia; per l'economia dei lavori di quest'Aula non sto a citarli, anche perché alcuni sono

nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza due ulteriori unità. Mi riferisco, in primo luogo, all'unità informativa scommesse sportive, con funzione di monitoraggio e analisi delle informazioni fornite dagli organismi preposti alla gestione delle manifestazioni sportive, per la conseguente proposta di mirate strategie preventive e repressive delle scommesse illegali e di rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia

con funzione di impulso e di raccordo dell'attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione del crimine organizzato nel mondo sportivo. Si tratta di risposte concrete tese

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». In sintesi, viene sancito che i soggetti che intendono esercitare un'attività nell'ambito delle scommesse devono ottenere una concessione, rilasciata dall'amministrazione finanziaria,

Numerose sentenze, sia dei giudici nazionali che della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno confermato la validità del regime del cosiddetto doppio binario (preventiva concessione o autorizzazione e successiva licenza di polizia) che non risulta in contrasto con il principio della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, senza considerare che il settore dell'attività di azzardo, che implica una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse è tra i cosiddetti settori esclusi dalla direttiva europea La proposta di modifica appare opportuna laddove stabilisce che l'intermediario, operante sul territorio nazionale, produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea per i necessari controlli, finalizzati al contrasto alla criminalità.

Anche l'Atto Senato n. 2714, per le ragioni appena espresse, si potrebbe opportunamente modificare. Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di scommesse,

Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in merito al ripetersi a Castellammare di Stabia di inquietanti episodi - uno, in particolare, molto grave che dimostrano la pervicace presenza sul territorio della criminalità organizzata e quanto siano pericolosi e sprezzanti i suoi metodi. Il 1° ottobre scorso, il quotidiano locale "Metropolis", che tira numerose copie ed è molto letto in varie aree della provincia di Napoli, è stato fatto oggetto di gravi intimidazioni:

e davvero molto forti. La camorra, battuta sempre più spesso dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, delegittimata anche nel giudizio di gran parte del popolo campano, continua ad alzare la testa. Abbiamo chiesto - e questa mattina intervengo in quest'Aula un intervento con prontezza per accertare la natura di tali episodi, i mandanti e gli esecutori. Inoltre, signor Presidente, se mi permette, invitare il Governo, ed anche il Parlamento, a trovare strumenti e azioni che diffondano la cultura della legalità e modelli positivi sui nostri territori. Signor Presidente, forse alcuni senatori avranno notato che davanti a Palazzo Montecitorio vi è una tenda con qualcuno che - si legge da

vi sarà un'ulteriore manifestazione dove si annuncia la partecipazione di un migliaio di persone per intavolare una discussione tra pari con i parlamentari. settimana prossima (per chi fosse a Roma nella pausa tra i lavori della mattina e quelli del pomeriggio), siamo tutti invitati ad andare ad ascoltare le ragioni di queste persone, che ci sono state fatte pervenire dal signor Stefano Sacconi.

di grande importanza nell'epoca della Rete, cioè la sospensione dell'attività di Wikipedia (o Wikipedìa: esistono diverse scuole di pensiero sull'accento) come come misura preventiva rispetto alla conclamata approvazione, temuta nel mondo della Rete, del disegno di legge sulle intercettazioni che, oltre al resto, reca un punto specifico

evoluzione ed in continuo rinnovamento, si rischierebbe sostanzialmente di creare una sorta di percorso accidentato, fino alla chiusura. Infatti, se qualcuno si mettesse d'impegno a chiedere una rettifica con tanto di pena, una struttura come Wikipedia non potrebbe più vivere. Pertanto l'attenzione è da porre su un tema di una delicatezza assoluta, che tra l'altro rischia di fare dell'Italia un Paese repressore della Rete, come la Cina o l'Iran.

Grazie,